finanziaria 2010)». Detto parere sara pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta odierna. Tenuto conto del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2010, ai sensi dell’articolo 126, comma 3, del Regolamento, preso atto della posizione del Governo, comunico che il disegno di legge finanziaria appare, nel complesso, in linea con le prescrizioni dell’articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, tra cui da ultima la legge n. 208 del 1999. Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 126, comma 4, del Regolamento, la Presidenza dichiara che il disegno di legge finanziaria non reca disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente, in base ai presupposti e alle interpretazioni fornite dalla Commissione bilancio. Deferisco pertanto i disegni di legge nn. 1790 (legge finanziaria per il 2010) e 1791 (bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012) alla 5ª Commissione, in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.